L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Comunico che in data 2 agosto è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (741). Il provvedimento è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 6a e 11a,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

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che siamo oggi chiamati ad esaminare è volto alla conversione in legge di un decreto legge, recante proroga di termini di disposizioni legislative. Il provvedimento, come di consueto, è stato necessario per disporre la proroga di termini di imminente scadenza, con l'obiettivo di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'operatività di fondi, anche a sostegno di investimenti, nonché per assicurare il completamento delle operazioni di trasformazioni societarie e di conclusione degli accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo. Passo ora, brevemente, all'illustrazione dei contenuti del decreto. Come sapete, il nostro Regolamento prevede che in Aula il testo sottoposto all'esame dei parlamentari sia quello originario. Quindi, partendo dal testo del Governo, è opportuno dare conto dei principali contenuti. Il provvedimento si compone di 14 articoli. L'articolo 1 reca proroga di termini in materia di enti territoriali. In particolare, il comma 1 ha ad oggetto i criteri di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio per Province e Città metropolitane. Al comma 2, la disposizione è finalizzata a individuare un'unica giornata nella quale si svolgeranno le elezioni dei presidenti di Provincia e dei consiglieri provinciali, il cui mandato viene a scadere entro il 31 il 31 ottobre 2018,

Il comma 1 prevede la proroga di termini in materia di programmi di edilizia scolastica, mentre il comma 2 proroga i termini in materia di salvamento acquatico. La disposizione contenuta nel comma 3 interviene, invece, in materia di obbligatorietà della patente nautica. L'articolo 5 ha ad oggetto la proroga di termini in materia di politiche sociali. In particolare, si proroga il termine di entrata in vigore della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) precompilata,

Il comma 3 proroga il termine relativo alle scuole italiane all'estero, consentendo il regolare avvio dell'anno scolastico 2018-2019 nel sistema della formazione italiana nel mondo. L'articolo 7 proroga i termini in materia di cultura. In particolare, si prevede espressamente l'estensione del beneficio del «*bonus* cultura» per l'anno 2018.

agli investimenti privati nelle strutture ospedaliere in Sardegna. Con l'articolo 9 sono prorogati i termini in materia di eventi sismici. Il comma 1 ha ad oggetto il recupero di aiuti relativi agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo, mentre il comma 2 ha ad oggetto il riparto del Fondo di solidarietà comunale nei Comuni del cratere Emilia-Romagna, colpiti dal sisma nel 2012, e del cratere dell'Aquila, per il sisma del 2009. L'articolo 10 ha ad oggetto la proroga di termini in materia di sport. L'articolo 11 reca proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi. L'articolo 12, al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni italiane, già finanziate con l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, Il rifinanziamento del Fondo è urgente e necessario al fine di evitare la sospensione dell'operatività dovuta all'attuale assenza di disponibilità per nuove Com'è noto, il Fondo è destinato all'erogazione di contributi in conto interessi a supporto di finanziamenti *export* (tramite operazioni di credito acquirente e credito fornitore) e di finanziamenti per l'internazionalizzazione. L'articolo 13 contiene una proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese. Infine, l'articolo 14 reca la disposizione concernente l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel corso dei lavori della Commissione affari costituzionali, che sono stati intensi a motivo del poco tempo a disposizione, sono stati affrontati molti temi, corrispondenti alle numerose proposte di emendamenti pervenute pressoché da tutti i Gruppi presenti in quest'Aula. Ci siamo confrontati e abbiamo valutato con attenzione e rigore moltissime questioni. Diversi emendamenti sono stati approvati e saranno ora sottoposti al voto dell'Assemblea, come da Regolamento, in qualità di emendamenti proposti dalla Commissione. Altri sono stati respinti; altri ancora sono stati dichiarati improponibili per estraneità con l'oggetto del decreto o inammissibili per difetto di copertura finanziaria. Cercherò, brevemente, di fare un quadro di insieme delle principali innovazioni scaturite dal lavoro della Commissione, pur consapevole che le proposte approvate sono molteplici e richiederebbero un'illustrazione ben più ricca e ampia di quella che, dati i tempi ristretti, possiamo concederci. In particolare, al primo articolo è stato approvato un emendamento in tema di elezioni per i Presidenti di Provincia, che si terranno il prossimo 31 ottobre. In occasione di tale tornata elettorale è ora previsto che, in deroga ad una disposizione della legge Delrio, siano eleggibili i sindaci il cui mandato scada non oltre dodici mesi dalla data della votazione. Sempre all'articolo 1 è stato approvato un emendamento in materia di procedura di controllo, di cui al comma 7 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Altro emendamento all'articolo 1 è quello che proroga di un ulteriore anno il termine entro cui effettuare le alienazioni relative alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche dopo opportuna ricognizione. È stato poi approvato un articolo 1-*bis*, recante proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali. All'articolo 2, in tema di giustizia, sono stati approvati diversi emendamenti, in tema di proroga del ripristino delle sezioni distaccate dei tribunali di Ischia, Lipari e Portoferraio. Sempre all'articolo 2, è stato approvato un emendamento che aumenta da cinque a sette anni i tempi di proroga per l'entrata in vigore delle nuove norme concernenti l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. All'articolo 3, si segnala in particolare un emendamento che proroga al 2020 l'entrata in vigore del libero mercato nei settori dell'energia elettrica e del gas per i consumatori finali. All'articolo 4 sono stati approvati emendamenti in tema di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane. Dopo l'articolo 4 è stato inserito un articolo 4-*bis*, recante proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali. All'articolo 6 è stato approvato, in particolare, un emendamento che proroga i termini entro cui gli edifici scolastici devono procedere all'adeguamento alla normativa antincendio. Sempre all'articolo 6 sono stati approvati alcuni emendamenti che differiscono all'anno scolastico 2018-2019 l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73. All'articolo 8, in tema di sanità, sono stati approvati alcuni emendamenti in tema di sigarette elettroniche e di medicinali omeopatici. All'articolo 9 sono stati approvati emendamenti che riducono o annullano i tagli operati negli anni passati al Fondo di solidarietà comunale. All'articolo 10, è stato approvato un emendamento in tema di adeguamento dell'ACI alle disposizioni di cui al recente decreto legislativo in tema di società partecipate. All'articolo 11 sono stati approvati degli emendamenti aggiuntivi in tema di sospensione della quota capitale dei mutui e finanziamenti e in materia di iscrizione nel nel registro delle imprese dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio. All'articolo 13, infine, sono stati approvati diversi emendamenti, tra cui uno in tema di spazi finanziari per le Regioni e due recanti proroga di termini in materia di Libro unico del lavoro telematico. *(Brusio).*

leggerò una parte della relazione che abbiamo già depositato agli atti, aggiungendo qualche elemento e riservandomi poi in sede di replica di fare alcuni approfondimenti anche in funzione di quella che

Chiaramente, le esigenze di tempo hanno in qualche modo consigliato alla maggioranza di procedere senza alcun intervento che ci desse indicazioni sulle volontà politiche presenti dietro ai provvedimenti contenuti all'interno del milleproroghe,

Chiaramente, l'uso dello strumento del decreto ha costretto la Commissione ad esaminare il testo con termini molto brevi, limitando enormemente la possibilità di sviluppare in Commissione un dibattito approfondito sul senso e la funzionalità delle modifiche proposte. L'istruttoria legislativa in Commissione ne esce così mortificata e fortemente limitata. Stupisce come le forze politiche dell'attuale maggioranza, che avevano promesso, anche aderendo alla riforma del Regolamento del Senato, una rinnovata centralità dell'attività delle Commissioni nel quadro di una ritrovata centralità dell'istituzione parlamentare nell'esercizio della funzione legislativa,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 Nell'esaminare il decreto-legge emergono, inoltre, rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento, per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso dello strumento del decreto-legge indispensabili per il suo legittimo utilizzo. Non è, infatti, sufficiente la mera dichiarazione di necessità ed urgenza per giustificare l'adozione di un decreto-legge se, come nel provvedimento in esame, il contenuto del decreto risulta carente dei requisiti prescritti dall'articolo 77 della Costituzione. Richiamo incidentalmente la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, che ha chiaramente affermato che i cosiddetti decreti milleproroghe che, con cadenza ormai annuale (qui c'è un ulteriore elemento di novità, perché questo è un decreto milleproroghe di mezza estate,

vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere incidere su situazioni esistenti, pur attinenti a oggetti e materie diversi, che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Ove le discipline estranee alla *ratio* unitaria del decreto-legge presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti a loro volta eterogenei. Tale ultimo caso riguarda, con tutta evidenza, il presente decreto-legge.

la garanzia della continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'operatività di fondi a fini di sostegno agli investimenti; dall'altro la necessità di assicurare il completamento delle operazioni di trasformazioni societarie e di conclusione degli accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo. cooperativo. L'eterogeneità dei contenuti è d'altronde cresciuta in sede di esame parlamentare; gli argomenti affrontati sono, se possibile, stati ampliati. Gli emendamenti approvati sono stati infatti numerosi ed eterogenei, ed hanno ulteriormente complicato un quadro in cui è stata dimenticata anche la minima ratio unitaria tipica del cosiddetto decreto-milleproroghe, quella di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo Un esempio che vale per tutti e che evidenzia l'intento di ampliare gli spazi di intervento del decreto ben oltre quanto sarebbe possibile: l'approvazione di un emendamento che procede a rimodulare gli spazi finanziari delle Regioni rispetto a quanto precedentemente previsto, senza oltretutto oltretutto rispettare le consuete procedure di consultazione degli enti locali attraverso la Conferenza delle Regioni. Sul merito stesso del provvedimento emergono forti perplessità. L'articolo 1, comma 2, fissa al 31 ottobre 2018 la data per lo svolgimento delle elezioni provinciali e proroga il mandato dei Presidenti di Provincia e dei consiglieri provinciali in scadenza fino a tale data; prevede inoltre che, in tale quadro, abbiano luogo contestualmente le elezioni del rispettivo Consiglio provinciale o Presidente di Provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018. La disposizione in esame non tiene conto che ad oggi, le scadenze dei mandati provinciali sono le seguenti: 47 presidenti di Provincia scadono entro il mese di ottobre 2018, 12 Consigli provinciali entro il 31 ottobre 2018, 15 Consigli entro il 31 dicembre 2018, 43 consigli entro il gennaio 2019. non è realizzabile nella data del 31 ottobre, perché la maggior parte delle province (43) delle Regioni a statuto ordinario, in base alla disposizione introdotta, sarà costretta a convocare le elezioni per il rinnovo degli organi

di candidarsi a Presidente della Provincia. La previsione dell'*election day* al 31 ottobre 2018 per le 15 province i cui consigli scadano entro il 31 dicembre 2018 comporta una interruzione anticipata del mandato che suscita gravi dubbi di costituzionalità, soprattutto perché esso non è giustificato da un più complessivo intervento di revisione della legge n. 56 del 2014. Tale situazione conferma Tale situazione conferma pertanto la necessità di un intervento legislativo che superi l'attuale precarietà dell'assetto del governo provinciale per dare una prospettiva certa di riassetto della disciplina in materia e agli attuali organi provinciali che svolgono funzioni di rilievo nel contesto economico e sociale nei loro territori

Mi avvio a concludere, citando sinteticamente altri punti che poi nella discussione generale verranno affrontati in modo più preciso dai colleghi del Partito Democratico, perché ci sono alcuni temi che gettano ulteriormente nell'incertezza il Paese su alcune questioni di assoluta importanza. Ancora una volta si è mancato di intervenire sulle questioni legate al terremoto e ai sismi del Centro Italia, e non solo, ma il Governo in Commissione ha dato ulteriori assicurazioni sui prossimi interventi nella legge di bilancio (vedremo se sarà così). se sarà così). È stata prorogata tutta la normativa legata alle intercettazioni. Sui vaccini, che è una materia assolutamente sensibile per tutto il Paese ed è legata alla sicurezza delle nostre famiglie,

Ma chi subisce le conseguenze di questo dilazionamento dei tempi? Il Paese. Pertanto, noi siamo qui anche per sottolineare questi aspetti e cercare di dare il nostro contributo.

di discussione generale sul decreto-legge milleproroghe. È dal 2005 che questo malvezzo della politica italiana viene perpetrato da vari Governi. Ricordo quando coloro che oggi siedono in maggioranza strillavano dai banchi dell'allora opposizione contro il milleproroghe dicendo che loro non ne avrebbero mai fatti. Oggi ci ritroviamo con un milleproroghe presentato dal cosiddetto Governo giallo-verde; un milleproroghe che peraltro ha visto anche un dialogo pressoché nullo con il resto del Parlamento: un milleproroghe che di fatto non ha colto il dialogo e il confronto con le opposizioni. Questa è una constatazione che certamente non depone a favore dei buoni propositi che dal Parlamento, negli anni passati, si erano manifestati in vista di un miglioramento dell'attività parlamentare. Comunque, entrando nel merito, tralasciando un milleproroghe che, come abbiamo visto, nei 14 articoli che lo caratterizzano salta dalle intercettazioni alle ricette veterinarie, possiamo notare come il *focus*, l'elemento forse più strutturale di tale decreto-legge, sul quale vorrei intrattenermi, sia la riforma del credito cooperativo, vale a dire la riforma della riforma Renzi-Padoan. Quella riforma che ha prima inciso negativamente sulle banche popolari e che avrebbe potuto - uso il condizionale incidere molto pesantemente sul credito cooperativo: incidere cioè molto pesantemente su una peculiarità del nostro sistema bancario, cioè il credito cooperativo. Quel credito che nella mutualità e nella territorialità esprime la sua caratterizzazione, che gli permette di rispondere alla particolarità del nostro sistema impresa e alla particolarità del nostro territorio. Chi vive nelle periferie di questo Paese, nelle valli (come me che provengo dal Trentino), sa che funzione hanno svolto e svolgono le casse rurali, il credito cooperativo, quelle banche che hanno i loro sportelli anche anche nelle cittadine e nei «paesoni» più sperduti del nostro territorio; quelle banche che permettono alle nostre imprese di avere comunque, a poca distanza dalle loro aziende

Se non ci fosse il credito cooperativo, come dimostrano i fatti, le banche cosiddette di interesse nazionale, le grandi banche, i due grandi gruppi che oggi sono rimasti nel nostro Paese, avrebbero, come hanno fatto, abbandonato i territori periferici. Noi non vogliamo che, nell'ottica della speculazione e dell'interesse finanziario, anche il sistema cooperativo debba, di fatto, allontanarsi dalle esigenze peculiari del nostro territorio. Ebbene, se la riforma Renzi-Padoan, se la riforma del credito cooperativo fosse rimasta tale o rimanesse tale, con con una capitalizzazione minima delle BCC nella capogruppo del 51 per cento, come era nelle ipotesi iniziali, sicuramente si sarebbero messe a rischio a breve la mutualità e la territorialità del credito cooperativo. Apprezziamo quindi, esprimendo un parere sicuramente favorevole, che il Governo abbia accolto la proposta che io, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia e in sede di audizione del ministro Tria, feci, chiedendo di elevare la capitalizzazione minima del 51 per cento ad almeno il 60 per cento. Questa non sarà una sicurezza, ma perlomeno blinda, in un certo qual modo, il patrimonio delle capofila, che resterà obbligatoriamente nelle mani delle casse rurali per almeno il 60 per cento. Ci auguriamo che questa strada venga ulteriormente migliorata dal Governo, nella moratoria di 180 giorni che prevede il decreto-legge, affinché si si renda più forte e strutturale la patrimonializzazione delle casse centrali da parte delle banche di credito cooperativo. Apprezziamo anche - e pure su questo chiediamo al Governo di essere ancora più incisivo e blindato e blindato - che sia stato previsto che la patrimonializzazione della capofila possa essere modificata solamente con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e non più con un semplice decreto ministeriale.

alternative per evitare che i capitali finanziari possano di fatto governare il sistema del credito cooperativo.

e ovvie dell'alta finanza, la possibilità di incidere sulle finalità mutualistiche, territoriali e speciali del credito cooperativo. Apprezziamo anche che sia stata elevata, nella *governance* delle casse centrali di ICCREA, alla metà più due la presenza obbligatoria dei consiglieri di amministrazione.

oggi ancora, in virtù della riforma in essere, in mano alle capogruppo, possa essere quanto più limitata. Vice ministro Garavaglia, signori del Governo, vi chiedo con forza di adoperarvi affinché le singole casse rurali, soprattutto quando la loro solidità patrimoniale lo permetta, possano avere quell'autonomia negli organi

una funzione ovviamente più speculativa e volta al profitto), possa immediatamente governare le singole

delle caratteristiche delle singole banche aderenti: infatti, se le singole banche sono più virtuose, ritengo che la capofila potrebbe avere anche dimensioni diverse. *(Applausi dal

si sta facendo tra luglio e agosto, in periodo preferiale (ma, magari, ci sarà l'intendimento di utilizzarne un altro verso fine anno).

evidentemente erano pretestuose. Era semplicemente la consueta accusa che veniva rivolta, in particolare, al Partito Democratico e comunque alla maggioranza della scorsa legislatura, dicendo che si voleva mettere il bavaglio al diritto all'informazione, che si voleva impedire che i cittadini conoscessero le conversazioni dei politici. Tutto questo significa solo due cose: cose: o il Ministro non conosceva il contenuto della riforma oppure tutte queste motivazioni erano strumentali. Come strumentali sono le motivazioni che vengono riportate nella relazione introduttiva a questo provvedimento per giustificare la proroga. In verità, il decreto milleproroghe,

sa che aveva ad oggetto il ruolo delle intercettazioni come fondamentale strumento di indagine, che creava un giusto equilibrio tra la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e, conseguentemente, l'equilibrio con il diritto all'informazione.

e ha obiettivi differenti da quelli denunciati dall'attuale maggioranza di Governo ed in particolare dal Ministro della giustizia. Si è introdotto infatti il reato di diffusione, di ripresa e registrazione di comunicazioni fraudolente per evitare che le intercettazioni vengano usate strumentalmente per denigrare magari anche qualcuno che non c'entra nulla con le indagini. Si è introdotta una maggiore tutela della riservatezza nelle comunicazioni tra difensore e assistito. Si tratta della salvaguardia di un elementare diritto di difesa: viviamo in un mondo di civiltà giuridica

vuole prorogare l'entrata in vigore di una norma di civiltà giuridica, che porta finalmente a sistema il giusto equilibrio tra il diritto di difesa e il diritto all'informazione, che tutela maggiormente tutti i cittadini e non la classe politica, che non c'entra nulla perché è trattata alla stregua di tutti i cittadini.

altrimenti il Governo ci spieghi le motivazioni di questa proroga.

Delrio (ribattezzata dagli amministratori locali «legge delirio»), ha rappresentato un esempio di psichiatria legislativa.

scritte soltanto nell'ottica pregiudiziale che il *referendum* costituzionale del dicembre del 2016 poteva trovare solo un giudizio di accoglimento da parte del

la dignità delle Province previste dalla Costituzione: ci troviamo al cospetto di un livello istituzionale che è stato completamente distrutto,

soprattutto nelle realtà di periferia della nostra Nazione, che sappiamo essere innanzitutto composta da Province, con migliaia di chilometri di strade provinciali abbandonate a se stesse, che non ricevono un intervento di manutenzione ordinaria da oltre quattro anni. Lo stesso ragionamento vale per le scuole medie superiori, con tantissimi operatori e alunni che corrono rischi gravissimi per la propria sicurezza. Delrio ha discriminato anche i dipendenti delle Province, ovvero il loro capitale umano, che è stato costretto a procedure di mobilità e ha corso anche il teorico rischio di licenziamento, pur trattandosi di dipendenti pubblici. I cittadini sono stati espropriati dal voto: c'è una politica che genera un altro livello politico, senza peraltro essere poi nella condizione di produrre risultati.

con la possibilità teorica anche di creare quella che viene definita un'anatra zoppa, con un presidente espressione di una parte politica e una maggioranza in Consiglio espressione dell'altra parte politica. I bilanci sono stati portati in maniera scientifica al dissesto: un dissesto di Stato, rispetto al quale, anche nei casi in cui non si riescano ad approvare,

le contraddizioni enormi e i guasti funzionali che ha prodotto la legge Delrio. Con la norma di proroga nostro esame, sembra che passiamo dalla psichiatria legislativa, alla legislazione creativa, perché immaginare di porre il termine di proroga al 31 ottobre 2018 significa ignorare che non per tutte le 47 presidenze, che saranno scadute a quel termine,

che oggi dovrebbero fare soltanto programmazione, invece fanno molta gestione, e i Comuni sono abbandonati al loro destino, soprattutto i più piccoli, i capoluoghi di provincia sono spesso vittime dei comportamenti da satrapi di Provincia di molti sindaci. Non è giusto che i cittadini paghino le conseguenze di scelte scriteriate, perché quelli delle realtà dei Comuni più piccoli pagano le stesse identiche tasse di coloro che vivono nelle realtà metropolitane o nei Comuni più grandi e hanno diritto ad avere gli stessi, identici servizi. Senza l'ente di governo in area vasta questa possibilità è assolutamente preclusa. Sanno bene tutti coloro che in questa Assemblea vengono da un'esperienza da amministratori locali, da assessori provinciali e da presidenti delle Province, cosa ha rappresentato la legge Delrio. Torno all'argomento della proroga, perché abbiamo presentato una proposta emendativa anche nell'auspicio che uno slittamento al 31 gennaio 2019 possa rappresentare un momento di riflessione all'interno del Parlamento, per tornare al suffragio universale. La guida delle istituzioni deve essere decisa dai cittadini. Questa proroga addirittura prevede la possibilità di sciogliere anticipatamente i Consigli rispetto alla data del presidente. Io conoscevo l'istituto della *prorogatio*, non quello della "*anticipatio*", che genererebbe certamente certamente un caso di incostituzionalità di questa norma. Concludo, signor Presidente, con un passaggio sull'articolo 10, che riguarda le Universiadi. Ho avuto modo in audizione di manifestare al sottosegretario Giorgetti tutte le mie perplessità rispetto ai ritardi relativi a questo importante evento, che sarà una vetrina internazionale per la Campania e per l'Italia. Rischiamo di fare una figuraccia, per la lite permanente e per l'irresponsabilità estrema del presidente della Regione Campania De Luca e del sindaco di Napoli De Magistris. Mancano dieci mesi alla celebrazione dell'evento e non è pronto assolutamente nulla, nulla, dalle strutture che devono ospitare gli eventi fino alla scelta del villaggio dove ubicare gli atleti. Mi sarei aspettato dal Governo non una scelta pilatesca, ma che prendesse in mano le operazioni, per fare in modo che i campani e l'Italia non ricevano l'umiliazione per il litigio di due uomini, che denota...

Signor Presidente, senatrici e senatori, membri del Governo, il mio intervento si concentra essenzialmente sull'articolo 2 di questo decreto-legge, in modo particolare sul comma 1, per ragioni completamente opposte a quelle prima riferite dal senatore Cucca del PD, il quale sostiene, dal suo punto di vista, l'accelerazione dell'entrata in vigore dell'attuazione di una norma di modifica della disciplina del sistema delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Bene, la posizione di Forza Italia è stata di contrarietà allora a quella riforma, perché perché si è trattato di una riforma assolutamente insufficiente, non in grado di assicurare il diritto di difesa, che ne veniva compromesso, e soprattutto non in grado di assicurare un momento centrale nella vita del nostro processo, cioè la segretezza delle indagini. È cosa ormai nota ed è una prassi assolutamente consolidata il corto circuito mediatico-giudiziario al quale siamo stati abituati e quasi mitridatizzati, per cui oggi ci è assolutamente indifferente anche convinti che esista la retroattività della norma penale. Quest'Aula ha avuto

perché non potevamo accogliere alcuni princìpi contenuti nella cosiddetta riforma della disciplina delle intercettazioni. Già allora, al momento dell'esame dello schema del decreto legislativo n. 216 del 2017, attuativo della delega, in Commissione giustizia la posizione di Forza Italia è stata chiara: violazione e forte compressione del diritto di difesa,

non chiarezza della novella dell'articolo 293 dello stesso codice. Perplessità che allora furono fatte proprie da molti procuratori, anzi dai procuratori delle maggiori città italiane perché quella riforma, che il PD allora volle a tutti i costi, in realtà si regge su un assunto per noi assolutamente non accoglibile, cioè quello secondo il quale sono gli avvocati i principali responsabili delle fughe di notizie durante la fase delle indagini preliminari. Ciò non è vero, o può esserlo solo minimamente in quanto la divulgazione dell'informazione

Siamo poi certi, riguardo all'altro dubbio che abbiamo sollevato, che l'applicazione dei nuovi dispositivi captatori informatici, così come previsto e regolamentato, sia immune da vizi e da abusi. Bene: noi, ripeto, eravamo contrari perché abbiamo ritenuto la riforma Orlando assolutamente insufficiente. Vorrei ricordare le parole di un magistrato, a volte scomodo ma sicuramente acuto nelle sue osservazioni, pronunciate allorquando fu approvata la riforma. Mi riferisco al dottor Nordio che ha affermato che la riforma costituisce il massimo degli sforzi consentiti con il minimo dei risultati perseguiti. L'unica cosa che avreste dovuto fare e non avete fatto è dare attuazione ad un codice. Le intercettazioni sono mezzi di ricerca della prova, non sono mezzi di prova. Le telefonate non solo delle prove. Voi avete consentito che il Parlamento perdesse tempo nell'attuazione di princìpi fondamentali del nostro ordinamento. Gli amici della Lega Nord spesso citano, giustamente,

vi vedremo allora all'opera non solo nella richiesta di proroga di un atto che per noi non è prorogabile, ma nel merito della riforma delle intercettazioni e nel far sì

Signor Presidente, intervengo sull'articolo 2 di questo provvedimento in materia di giustizia, quale componente della Commissione giustizia, per esprimere la soddisfazione mia e del collega Stancanelli

della nuova disciplina in materia di esame per la professione di avvocato. Come sapete, attualmente i candidati si sono preparati tenendo presente una disciplina che consente l'utilizzo dei codici commentati. Sarebbe stato assurdo, dopo che i candidati si erano preparati sapendo di poter utilizzare questi codici, vietarglielo. Quindi siamo soddisfatti dell'accoglimento di questo emendamento. Siamo invece perplessi e non comprendiamo le ragioni per cui siano stati respinti altri nostri emendamenti in materia di giudice onorario di pace e in materia di avvocati cassazionisti, perché venivano incontro a richieste più che ragionevoli avanzate da queste stesse categorie. Auspichiamo che l'Aula possa invece prendere in esame con un parere favorevole questi nostri emendamenti. Approfitto del tempo a mia disposizione, signor Presidente, sempre in materia di giustizia, per esprimere la soddisfazione del mio Gruppo per il brillante risultato conseguito dalle Forze dell'ordine che hanno ottenuto un rapido accertamento dei responsabili del grave atto di lesioni a carico della nostra atleta Daisy la quale rischia, appunto, di perdere anche un'importante occasione agonistica a causa del trauma riportato. A quest'atleta va l'abbraccio di tutto il Gruppo Fratelli d'Italia. E mi permetto di esprimere anche la soddisfazione per il fatto che,

Al di là della polemica, ci uniamo alla soddisfazione per l'azione delle Forze dell'ordine. È iscritto a parlare il senatore Comincini.

ai rinvii che riguardano la legge Delrio, non senza aver prima precisato ai colleghi che sono già intervenuti e a tutta l'Assemblea la riforma Delrio non ha previsto tagli alle risorse degli enti territoriali. Bisogna saper scindere gli aspetti della costruzione della *governance*, che la legge Delrio ha disegnato all'interno di una visione di sistema, che abbiamo avuto, da aspetti di bilancio: si tratta di due questioni estremamente differenti e diversificate. Ieri il vice presidente del Consiglio Di Maio, rispondendo ad un'interrogazione, ha voluto sottolineare ulteriormente in quest'Aula che il Governo intende ridurre gli sprechi,

per le amministrazioni, perché, in alcuni casi, devono essere convocate nel giro di poche settimane due elezioni diverse. Ora, stanti le scadenze differenziate dei presidenti delle Province e del Consiglio, è evidente che quanto previsto non è realizzabile nella data del 31 ottobre, perché la maggior parte delle Province delle Regioni a statuto ordinario - ben 43 - in base alla disposizione introdotta, sarà costretta a convocare le elezioni per il rinnovo degli organi ad ottobre per il presidente della Provincia e a gennaio per il Consiglio provinciale, come dicevo poc'anzi, con un'evidente duplicazione di procedure e costi. Inoltre, la previsione dell'*election day* al 31 dicembre 2018, per le 15 Province i cui Consigli scadono entro il 31 dicembre 2018, comporta un'interruzione anticipata del mandato che ha suscitato in diversi soggetti e analisti anche dubbi di costituzionalità, soprattutto in mancanza di un intervento organico di revisione della legge n. 56 del 2014. La legge Delrio prevedeva una serie di misure nell'ipotesi - auspicata certamente dal Partito Democratico - che la riforma costituzionale sarebbe stata approvata dal *referendum* del dicembre 2016. Ciò non è avvenuto e non è stato ancora possibile intervenire nel ridisegnare l'assetto complessivo degli organismi territoriali dello Stato. In attesa che ciò avvenga, non è possibile pensare di spezzettare in questo modo le elezioni dei presidenti. Servirà unificare la data per agevolare il lavoro delle Province ed evitare sprechi di denaro pubblico nell'organizzazione di doppie elezioni per presidenti e Consiglio. Mi auguro che nel dibattito legato agli emendamenti ci possa essere spazio e ascolto da parte la maggioranza per accogliere quanto stiamo dicendo e che anche da altre parti è stato evidenziato. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, abbiamo già detto con chiarezza quali sono i tratti di incostituzionalità che secondo noi

c'è un cambiamento rispetto al passato: l'unico cambiamento è che si faranno due provvedimenti milleproroghe.

che c'è tra le elezioni dei presidenti dei Consigli provinciali e i Consigli provinciali. Non si può dare la responsabilità di questo alla legge Delrio, che pure secondo me è una legge che ha dimostrato drammatici limiti. È una scelta che ha voluto fare il Governo. Abbiamo anche cercato in Commissione di trovare una sintesi tra le diverse ipotesi, ma non è stato possibile neanche questo. Abbiamo cercato anche noi, come altri colleghi, di sostenere gli emendamenti dell'Unione delle Province: non è stato possibile. Francamente non ho nemmeno capito perché; forse ci sono ragioni

siamo di fronte a un problema serio e grave che riguarda l'assetto dei Comuni e delle Province.

È che in quest'Aula l'unico momento topico è quando c'è qualcosa che non dovrebbe essere in quest'Aula: questo è il problema. Detto questo, il vero problema è: quale strategia avete rispetto agli enti locali e alle Province? C'è un problema di risorse grande come una casa. C'è un problema di motivazione motivazione che riguarda il personale che lavora negli enti locali, perché non possiamo continuare a parlare dei cartellini dei lavativi, quando l'attenzione non va a ladri e fannulloni.

tutto. Intervengo qui solo per sottolineare un punto. C'è un impegno del Governo al quale noi abbiamo dato fiducia: fatto che nella prossima legge di bilancio deve essere affrontato l'insieme dei temi che riguardano il centro Italia, L'Aquila, su cui c'è una grande urgenza - ricordo che il Governo si era impegnato a dare una risposta

Su questo sono indispensabili delle risposte. Noi continuiamo ad avere fiducia, ma poi occorrono i fatti. Un ultimo punto riguarda il tema dei vaccini.

di fare passi indietro. Mi sembra un atteggiamento ideologico. Anche per queste ragioni il nostro voto sarà contrario.

niente di tutto questo:

provvedimento, che è assolutamente blindato, chiuso, con uno stato d'animo della maggioranza impermeabile e anche un po' saccente. In poche parole, non si capisce che c'entra questo milleproroghe con l'urgenza che voi avete richiamato - poco fa il senatore Errani giustamente

nell'immediata vicinanza della pausa estiva, verrebbe naturale pensare che ci si sia messi in testa di fare qualcosa di positivo e tutto questo noi non lo abbiamo potuto verificare. Anzi, colleghi,

Per la seconda volta intervengo in Aula per mettere in risalto che ci sono pezzi d'Italia che aspettano di incontrare lo Stato con la S maiuscola; lo Stato che si fa vivo, si fa presente, risolve qualche problema, mette a posto qualche virgola nelle numerosissime regolamentazioni che accompagnano i privati cittadini e i tecnici impegnati nel processo della ricostruzione,

serissimo rischio di spopolamento. Quella gente ancora non ha visto iniziare la ricostruzione. Quella gente ancora è ospitata nelle casette di legno, in parte negli alberghi, a casa degli amici o con l'autonoma sistemazione. Qual

quelle benedette pratiche cominciano ad arrivare. Gli uffici che devono espletare le pratiche sono pieni di collaboratori che hanno contratti a tempo determinato, contratti atipici. Se non

sempre successo - a fare un nuovo milleproroghe che voi nelle scorse legislature contestavate dicendo che le proroghe dovevano essere eliminate. E qui invece lo fate come primo atto del vostro Governo, incapaci di fare politiche per le scelte dei cittadini. Seconda questione: abbiamo presentato un emendamento, a prima firma del collega Faraone, sulle disposizioni anticipate di trattamento per il fine vita. Altra grande ambiguità di questo Governo. La ministra Grillo ha usato parole importanti in questi giorni dicendo che per lei quella legge, che anche il partito del MoVimento 5 Stelle ha votato nella scorsa legislatura, deve essere attuata definitivamente. Noi abbiamo proposto una proroga per un termine che è già scaduto. Doveva essere fatto un decreto per le modalità della banca dati, ma nell'attesa che voi faceste il vostro contratto e formaste il vostro Governo, per fare questo decreto non c'è stato tempo. quindi una proroga ad ottobre, ma quell'emendamento è stato respinto. Forse perché la Lega, vostra alleata, non è d'accordo sul fine vita? Forse anche questo atto si vuole scompaginare? Abbiamo bisogno di chiarezza. Non è più il caso di dire tutto e il contrario di tutto sulla TAV, sui vaccini e su quel che riguarda il fine vita. L'ultima questione è la più rilevante. Facendo parte della Commissione sanità, mi unisco all'allarme lanciato ieri dai miei colleghi Dario Parrini e Simona Malpezzi in Commissione. Considero gravissimo il fatto che si sia prorogata di un anno la possibilità dell'obbligo vaccinale per i bambini che si vogliono iscrivere negli asili. È notizia di oggi di due bambine morte di pertosse in questo Paese. Credo che tutti voi vi dobbiate mettere una mano sulla coscienza. Mi auguro che dormirete

abbiamo sentito la ministra Grillo dire che voleva fare l'autocertificazione. È chiaro ed evidente a tutti che non si può modificare una norma con una circolare ministeriale.

State facendo un danno alla salute dei cittadini e dei più deboli. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Dovrete decidere, prima o poi, se volete governare questo Paese, seguire la scienza, ascoltare i medici, tutelare l'interesse dei cittadini o pensare alle *fake news* oppure alle scie chimiche.

e devo dare atto al Presidente di non aver in alcun modo soffocato il dibattito, che peraltro non è stato un dibattito, signor Presidente e onorevoli colleghi, ma un monologo. parlato infatti soltanto l'opposizione; credo che lo abbia fatto in maniera non ostruzionistica, ma mirata su alcune problematiche sensibili, sulle quali non c'è stato uno straccio di risposta. Noi ci siamo impegnati a dare delle motivazioni su alcuni punti essenziali *(Applausi dal Gruppo FI-BP e PD)*, ma non c'è stata una risposta né da parte della maggioranza e né da parte del Governo. Non mi sembra questo un modo corretto di portare avanti i nostri lavori. È vero che i colleghi della Lega, con i quali abbiamo governato, avevano già usufruito del sistema del milleproroghe. Mi meraviglio però moltissimo della facilità e della *nonchalance* con la quale anche il MoVimento 5 Stelle, che nella scorsa legislatura ha fatto un cavallo di battaglia l'impossibilità di ricorrere a strumenti che soffocano il dibattito parlamentare e fanno venire meno i diritti dei parlamentari, si sia subito assuefatto al clima del Governo e del potere. Anche il MoVimento 5 Stelle - benvenuto tra noi - utilizza così questo strumento,

Voglio soffermarmi su due o tre punti, signor Presidente, perché le problematiche e le criticità del milleproroghe - che poi è un 500 proroghe perché in effetti non utilizza tutto il termine - sono molteplici

ha emanato il provvedimento per mettersi al sicuro dalla scadenza di alcuni termini e di alcune prescrizioni. Questo non è un buon costume. Credo che le leggi vadano rispettate nei modi e nei termini stabiliti, senza assumere la consuetudine di rinviare, molte volte *sine die*, l'adempimento

siano rimasti completamente sordi alle richieste avanzate. Mi riferisco, signor Presidente, onorevoli colleghi, alla norma che stabilisce l'elezione delle Province al 31 ottobre 2018, per tutte quelle che sono scadute fino a quella data. E fin qui potrebbe non esserci alcun problema. Il problema nasce nel momento in cui con una norma e con effetto retroattivo si fa scadere anticipatamente il mandato elettorale di un organo costituzionale, ancorché di un ente di secondo grado.

proposta dell'opposizione di stabilire *l'election day*. Ci riempiamo sempre la bocca sull'*election day* e sulla necessità di ottimizzare le elezioni e tagliare le spese. Avevamo proposto di rinviare tutte le elezioni dei presidenti e dei consigli al 31 gennaio. Anche «Il Sole 24 Ore», che evidentemente non era presente ai lavori della Commissione questa mattina, oggi titola «*Election day* delle Province al 31 gennaio 2019». Evidentemente aveva fatto un atto di fede e di fiducia nei confronti della maggioranza e del Governo, che invece è stato tradito, perché

C'è stato un ricorso al Consiglio di Stato, che ha dato la sospensiva e ha fissato l'udienza di merito al 18 ottobre.

in società per azioni. Se il Consiglio di Stato dovesse non confermare la sospensiva e quindi dare ragione al legislatore, i crediti cooperativi si troverebbero ad avere un ristretto arco di tempo per adempiere agli obblighi di legge. Anche in questo caso non capiamo la *ratio* del diniego ad accettare siffatta riformulazione.

prevedendo la deroga per le scuole che frequentano i nostri figli, i ragazzi, dove occorre garantire sicurezza, e non avete accolto la richiesta proveniente dagli imprenditori turistici che chiedevano una proroga. Ma sappiamo quale sia l'attenzione che voi riservate a questo settore, visto che avete violato anche l'adempimento di un ordine del giorno con il quale vi eravate tutti impegnati a prorogare l'entrata in vigore della direttiva Bolkestein. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendendo in prestito il titolo di un film del 1976, «Vizi privati, pubbliche virtù», credo che questo Governo e questa maggioranza fino ad oggi abbiano mostrato più i loro vizi che le loro virtù e siamo soltanto all'inizio. Buon lavoro.

sicuramente, qualora capiterà un'altra volta, provvederò a posizionarmi nel posto giusto. Credo che la replica sia d'obbligo, perché la discussione generale è andata avanti sulla falsariga

milleproroghe è un provvedimento che ha le caratteristiche che abbiamo descritto in discussione.

è il tempo. Come si fa ad aggredire e attaccare gli elementi che strutturalmente impediscono di dare omogeneità al nostro Paese? Si fa con le riforme.

occasione. Occorre gradualità, i processi non sono istantanei, i cambiamenti non possono essere portati avanti in un secondo, bisogna costruire un percorso. La prospettiva quindi è data dalle riforme e, quando è toccato a noi, lo abbiamo fatto. Capisco

un contratto, che non c'è bisogno di farselo piacere: un contratto, dopo che lo si è firmato, è sottoscritto. Certe volte ascoltare alcuni interventi mi fa anche un po' tenerezza, perché contengono lo sforzo di motivare dal punto di vista

Nel decreto milleproroghe in esame si affronta il tema delle Province, in un modo anche abbastanza privo di prospettiva: si fanno delle modifiche, sono contenuti forse degli obiettivi non detti fino in fondo,

che tenete nel cassetto, e quindi le Province sono contenute in un altro pezzo di accordo; oppure dovete riscrivere meglio la clausola conclusiva di ogni contratto per quanto non contemplato dal presente contratto si fa come dice la Lega. Dico questo perché ci sono delle evidenti contraddizioni. Io sto cercando di sollecitare questa maggioranza a guardare a temi di prospettiva, di visione,

Due anni fa noi disponemmo la proroga, ma mettemmo in campo un piano nazionale di sostegno agli enti locali per finanziare per tre anni la messa a norma delle scuole.

il *gap* infrastrutturale che va colmato. Noi avevamo previsto 47 miliardi di euro per le opere pubbliche e infrastrutturali: oggi voi prendete tempo per fare delle valutazioni. Lo sappiamo: è su tutti i giornali la vostra discussione sulle valutazioni che dovete fare sulla necessità e sulle caratteristiche delle infrastrutture, ma le infrastrutture sono importanti, per dare competitività al nostro Paese. Voglio dunque ribadirlo in conclusione del mio intervento, perché si possono

la Presidenza, in conformità a quanto stabilito in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti già presentati in Commissione: 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.27, 1.30, 1.45, 1.46, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.91, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 2.26, 3.17, 3.19, 3.20, 4.22, 4.0.1, 5.8, 5.0.3,

8.11, 8.13, 9.10, 9.11, 9.24, 9.25, 9.33, 9.34, 9.43, 9.48, 9.52, 9.53, 9.82, 9.92, 9.97, 9.98, 9.99, 9.101, 9.102, 9.103, 9.0.1, 9.0.4, 11.11, 11.0.5, 1.11, 1.33, 1.34, 1.41, 1.42, 1.43, 1.50, 1.51, 1.52 e 11.7 (limitatamente alla lettera *b*), in quanto estranei all'oggetto del decreto-legge. Per le medesime ragioni la Presidenza dichiara improponibile anche il nuovo emendamento 5.0.300.

estremamente preoccupati per le notizie, sempre più precise e sempre più numerose, in merito agli attacchi *web*, frutto di manovre che al momento risultano estremamente oscure e torbide,

Quello che sappiamo fino a questo momento è sufficiente per indurci a chiedere a lei di rappresentare al Presidente del Consiglio la nostra convinzione che sia estremamente urgente la sua presenza in quest'Aula per riferire al Senato su cosa è a conoscenza del nostro Esecutivo, sulle iniziative che si intendono intraprendere e su ciò che si è deciso di mettere in campo per fare chiarezza su questa cosa estremamente grave. Come tutti hanno potuto leggere nei numerosi articoli usciti negli ultimi due giorni, la notizia relativa a questi attacchi è stata ricavata da un'indagine Si parla di decine e decine di profili falsi, di fabbricazione straniera, di origine russa, vicini agli apparati di sicurezza del Governo russo, siti che hanno diffuso attacchi delegittimanti, infamanti e gravemente intimidatori nei confronti del Capo dello Stato in un momento cruciale della vita politica nazionale. Sappiamo tutti, per i numerosi dibattiti che sono stati fatti in merito al potenziale distorsivo sul piano democratico della diffusione coordinata e organizzata di *fake news*, quanto queste pratiche, estremamente inquietanti e torbide, possano manomettere e inquinare la vita democratica di un Paese. Dobbiamo avere piena coscienza del pericolo che queste iniziative rappresentano e dobbiamo fare assoluta chiarezza. In altre sedi il mio partito ha chiesto che di questo si occupi il Copasir; è una richiesta che ovviamente noi sottoscriviamo. La collega Quartapelle ha chiesto che il Governo convochi immediatamente l'ambasciatore russo e anche questa è una richiesta che sottoscriviamo, perché il Capo dello Stato, che è la massima carica della Repubblica, non può difendersi da solo ed è necessario che il Governo dia immediatamente un segnale di grande attenzione alla gravità di quanto sta emergendo. *(Applausi dal Gruppo PD e poiché questa vicenda presenta implicazioni, sia di sicurezza nazionale che internazionale, credo che sia necessario che a riferirne in quest'Aula venga direttamente il presidente del Consiglio Conte. Sono sicuro che questa nostra richiesta sarà considerata con grande attenzione dalla Presidenza, che ringrazio anticipatamente. Aggiungo che noi non siamo sovranisti, non siamo sovranisti, ma vediamo che questa vicenda solleva questioni pesanti che hanno a che vedere con la salvaguardia e con l'integrità della sovranità nazionale dell'Italia: chi si definisce con grande autocompiacimento sovranista dovrebbe essere preoccupato, non quanto noi, ma persino più di noi.

indicando alcune scadenze che avevano necessità di essere prorogate e che abbiamo ritenuto dovessero essere poste all'attenzione

parlo solo di quelli riferiti all'articolo 1 - concernenti gli enti locali, i Comuni, le Province e tutto ciò che aveva comunque a che fare con l'andamento del regolare svolgimento degli anni scolastici, anche quanto fosse necessario e opportuno andare incontro ad alcune esigenze riguardanti il buon andamento e la buona amministrazione di alcuni Comuni importanti. Per questa ragione abbiamo inteso proporre

l'attuale assoluta assenza di finanziamenti pubblici e che vivono una situazione di gravissima decozione. Questi emendamenti non sono stati ritenuti utili dalla maggioranza, che li ha respinti, ma noi pensiamo che essere solidali ed avere attenzione nei confronti dei piccoli Comuni sia assolutamente necessario. abbiamo ritenuto fondamentale - e in questo abbiamo avuto accoglimento - ottenere una proroga sulle misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020, così come sollecitato, per la verità, dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani e questo sostanzialmente è stato accolto, successivamente, dalla 1a Commissione, che ha riformulato un proprio emendamento che ha comportato la possibilità di venire incontro a questa istanza, che c'è stata rivolta dall'ANCI. Abbiamo poi inteso affrontare un tema assolutamente urgente, che ci è stato sollecitato da un caso particolare, relativo al Comune di Catania, laddove all'indomani delle ultime elezioni locali tenutesi la scorsa primavera,

onde consentirle il tempo necessario per avviare un piano di riequilibrio rimodulato e riformulato in base al comma 888 dell'articolo in

affari costituzionali affinché questo emendamento fosse accolto. Poiché c'è stato un corto circuito che mi è sfuggito, non so se il presidente della Commissione Borghesi può

1.9, sulla questione delle Province, che è stata all'attenzione della Commissione e dell'Assemblea. Noi avevamo proposto una misura che ritenevamo estremamente ragionevole, che era quella di posticipare tutte le elezioni al 31 gennaio Ebbene, mi sento di esprimere con estrema chiarezza una questione che non riguarda ovviamente Forza Italia, ma lo debbo dire con la stessa semplicità con la quale ce lo siamo detti in Commissione ieri sera e stanotte: qui ci sono due elementi in campo, da una parte, il Partito Democratico che difende la possibilità di posticipare le elezioni delle Province e, dall'altra, la maggioranza o un pezzo di questa che difende la possibilità di anticiparle tutte al 31 ottobre, perché, entrambe legittime? Perché sono in scadenza le fondazioni bancarie. Ebbene, noi a questo giochetto non ci stiamo e di conseguenza, se ve la volete suonare e ve la volete cantare, per noi ve la potete anche ballare, perché su questo non siamo assolutamente d'accordo e a questi giochetti sulle banche - che mi sembra siano stati già una caratteristica della precedente legislatura, che non è andata poi particolarmente bene - riteniamo di non dover partecipare. Forza Italia è un'altra cosa e mi pare che ogni giorno emerga sempre di più.

per la predisposizione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, nonché a bloccare

che, rispetto a quel tempo, alcune emergenze relative alla sicurezza e all'immigrazione implichino la necessità di avere un organico maggiore e più forte. Con riferimento

salverebbe l'integrità delle prefetture e andrebbe a incidere soltanto su quegli incarichi speciali che nel frattempo sono maturati. Se così fosse e se ciò fosse confermato Governo, sarebbe già un risultato notevole, perché non verrebbero meno l'autorevolezza e la forza dello Stato in un momento che mi sembra

del Governo a dire qualcosa in proposito, avendo la disponibilità anche a ritirare, nel caso, l'emendamento. In caso contrario, mi accontenterò mi accontenterò del fatto che ci sia stato comunque uno stimolo affinché il problema della riorganizzazione sia preso in considerazione senza che l'apparato dello Stato, in particolare quello delle prefetture, ne abbia a soffrire. senatori Iannone Signor Presidente, illustrerò soltanto le ragioni dell'emendamento 1.4, perché gli altri emendamenti presentati in rappresentanza del Gruppo Fratelli d'Italia

Signor Presidente, mi rifaccio a quanto detto dal senatore Pagano, perché vi è un emendamento a mia firma, l'1.105, che è è uguale all'emendamento 1.106. Ieri, in Commissione affari costituzionali, il Presidente della Commissione ha proposto una riformulazione dell'emendamento e, per come ci era stato illustrato, avevamo dato il nostro assenso. Tuttavia, leggendo ora il testo, non mi pare che si raggiungano gli scopi che il mio emendamento vuole raggiungere. In pochissime parole, l'emendamento 1.105 tende a riaprire i termini per le amministrazioni che si sono insediate quest'anno e fissare il termine del 30 settembre per ripresentare un piano di riequilibrio, sospendendo eventuali decisioni della Corte dei conti.

senatrice De Petris

Il Ministro dell'interno ha recentemente dichiarato la sua volontà di istruire al più presto un percorso per modificare gli assetti delle Province e riformare gli enti locali. Credo che questo percorso avrebbe bisogno di tempo, invece il testo del milleproroghe anticipa le scadenze elettorali,

Troviamo incomprensibile questa scelta. Siamo d'accordo con l'Unione delle Province italiane che tale scelta dovrebbe essere rigettata e voteremo a favore di questi emendamenti per questa ragione. Signor Presidente, il comma 2 dell'articolo 1 apparentemente è virtuoso, perché stabilisce un *election day* per l'elezione dei Consigli provinciali;

per cui noi, con questo emendamento, accorciamo la durata della vita di un Consiglio, di un'istituzione garantita dalla Costituzione, di tre mesi, senza alcuna ragione evidente. È un precedente estremamente pericoloso, la cui *ratio* non è sicuramente riconducibile ad alcun tipo di ragionamento istituzionale o costituzionale. Prima il senatore Mallegni ha ricordato forse la ragione vera di questa anticipazione: voler procedere con una rinnovata *governance* ai rinnovi di fondazioni bancarie estremamente importanti. Trattare così la Costituzione, a scopi assolutamente incomprensibili e inaccettabili, è veramente molto pericoloso e costituisce un precedente che non avrei mai voluto veder apparire nell'Assemblea di questa istituzione così importante, quale è il Senato.

in dissenso dal Gruppo.

2018 di presentarsi, entro i dodici mesi, quali candidati alle Presidenze delle Province. Purtroppo ci siamo dimenticati che 4.000 degli 8.000 Comuni italiani votano nella tornata primaverile del 2019 e in alcune Province

Forse il Parlamento dovrebbe leggere queste realtà e metterle nelle condizioni di funzionare. Non faccio la nemesi storica della legge Delrio, ma a questo punto si valuti qual è la realtà

senatore Pagano

per chiarire e magari per aiutare lo svolgimento ordinato dei lavori: il Partito Democratico insiste sulle votazioni dei soli emendamenti che riguardano la tematica del terremoto. In tutti gli altri casi, dove c'è parere contrario ai sensi dell'articolo 81, noi non insistiamo per la votazione.

1.680 è stato ritirato.

Forse ho dimenticato di chiarirlo.

i senatori Segretari a controllare che le votazioni avvengano in modo regolare.

2.6 trattano del ripristino temporaneo delle sezioni distaccate insulari anche di Lipari e di Portoferraio.

desidero segnalare che la situazione dell'insularità sotto il profilo della giustizia va equiparata. Era stato prorogato il termine per la sezione distaccata di Ischia e l'emendamento 2.7 proponeva tale proroga anche per la sezione distaccata di Lipari e per la sezione distaccata di Portoferraio. Abbiamo apprezzato il fatto che la Commissione abbia fatto propri gli emendamenti e abbia sanato questa che sarebbe stata una disparità fra le situazioni identiche della giustizia nelle isole.

la possibilità di avere una sezione distaccata sarebbe stato veramente un grande guaio. Noi rivendichiamo in maniera forte questa modifica e crediamo di aver reso un servizio alla comunità dell'Elba.

La legge è entrata in vigore nel novembre scorso e gli organismi pagatori si sarebbero trovati chiaramente in crisi, perché più di un milione di certificazioni avrebbero dovuto essere gestite, creando problemi in termini di pagamenti

2.21, 2.22 e 2.23, che riguardano la magistratura onoraria e di pace. Abbiamo ritenuto di presentare questi emendamenti perché tutte le associazioni

dei magistrati onorari, tramite una completa modifica della recente "riforma Orlando", affrontando anche le questioni attinenti al trattamento ad essi spettante e alle coperture previdenziali ed assistenziali». Se questi nostri emendamenti non venissero approvati, questa riforma (considerata sia dagli interessati, che dagli amici che hanno sottoscritto il contratto di Governo penalizzante per la magistratura onoraria) noi ci troveremmo successivamente in grande difficoltà. Vorrei osservare che la tradizione italiana del giudice conciliatore, che poi si è trasformata in quella dei giudici onorari, ha reso tanta giustizia nei luoghi più sperduti del nostro Paese, del nostro Paese, a maggior ragione oggi che gli stessi magistrati ordinari dicono che senza l'attività, il sacrificio e la capacità

La relazione al comma 1 dell'articolo 2 recita: «Proroga del termine di applica di disposizioni in materia di intercettazioni», e si riferisce ad alcune questioni strutturali di risorse e di beni.

completamente la disciplina delle intercettazioni. Questo provvedimento, frutto di un lavoro molto approfondito che ha coinvolto non soltanto gli operatori di giustizia, ma il mondo del giornalismo, l'avvocatura, la magistratura l'università, tiene conto dell'importante e delicato equilibrio tra diritto alla riservatezza, ricerca della prova necessaria per assicurare i responsabili di reato e libertà libertà di informazione. Nulla di tutto questo sembra essere oggetto del rinvio che noi teoricamente dovremmo votare. Ci saremmo aspettati, se questo era l'oggetto, che il provvedimento effettivamente se ne facesse carico. Aggiungo Aggiungo che questa riforma delle intercettazioni prevede anche un importante potenziamento dello strumento di indagine sui reati di corruzione. con questo rinvio si intende rinviare molto in là nel tempo uno strumento più efficace e stringente per colpire il fenomeno della corruzione, sul quale a parole sembra sembra che ci si voglia molto scagliare? Oppure, invece, si vuole stravolgere un'importante riforma che affronta con molto equilibrio il tema della pubblicazione di quelle conversazioni e comunicazioni che non sono rilevanti per perseguire il reato? Vi chiedo quindi se siete sulla linea delle principali procure italiane, sulla base delle quali è stato forgiato e scritto il provvedimento. È un problema di come fare o se fare? Quali sono gli strumenti, al di là delle battute delle allusioni, che abbiamo ascoltato in questi ultimi giorni? Vogliamo evitare che le indagini si trasformino in un raccoglitore cieco e pigro di informazioni di qualsiasi tipo e natura, che non servono alla repressione dei reati e potenziare invece lo strumento di indagine? Il rinvio non è in alcun modo giustificato o argomentato, perché altrimenti sarebbe stato ristretto esattamente a problemi di struttura. Ci si sarebbe adoperati adoperati al riguardo. Tra l'altro, c'è stato un *iter* molto articolato; tutti questi argomenti dovrebbero essere conosciuti dal Governo e, in particolar modo, dal Ministro della giustizia che ha fatto parte della Commissione giustizia e partecipato alla stesura del provvedimento, seguendo tutte le tappe che lo hanno contraddistinto. In conclusione ci chiediamo quale sia l'impostazione, ma soprattutto quale sia quale sia l'idea sulle due importanti parole che echeggiano in questi giorni: sicurezza e libertà.

del consiglio di amministrazione della RAI in violazione di tutte le garanzie previste dall'ordinamento? È la pubblicazione indiscriminata di qualsiasi conversazione? È il combinato disposto sulla sicurezza di lasciare soli i cittadini di fronte ad di violenza e discriminazione, come quello preannunciato sull'abolizione della cosiddetta legge Mancino? Per noi sicurezza e libertà sono inscindibilmente legate e hanno un significato preciso che, ci pare, non coincida con il vostro.

che attualmente gli uffici non sono in grado di implementare l'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni. L'unica motivazione per noi è questa; non si può far entrare in vigore una disciplina nuova che non può trovare attuazione. Invitiamo pertanto il Governo e gli uffici del Ministero della giustizia a rendere possibile l'attuazione della nuova

detto che sembra non avere molto senso un elenco di specie invasive su un territorio così ampio, visto che è provato scientificamente che alcune specie sono invasive in un certo ecosistema e non in un altro e pertanto

la tempistica legata alla denuncia della detenzione di questi animali. Ricordiamo che il testo che stabiliva l'obbligo di denuncia è del 15 dicembre 2017

Ora, visto che la scadenza sarebbe stata al 15 di agosto, arriva improvvisamente una proroga di ben dodici mesi e mezzo. Poiché la denuncia comporta la compilazione di un modulo con l'aiuto del veterinario

molto colpevolmente tale articolo non comporta l'obbligo di denuncia per la detenzione di specie vegetali invasive. Ricordiamo che la quantità di miliardi di dollari persi a livello mondiale a livello mondiale per la diffusione spontanea, non voluta, o lo scambio di materiale vegetativo di propagazione (che siano rizomi, semi o talee) è enorme, quindi il Governo dovrebbe provvedere in tal senso a prevedere l'obbligo di denuncia anche per queste specie, anche perché c'è un'incongruenza: da una parte c'è l'obbligo di controllo e distruzione di queste specie invasive e, dall'altra, non c'è obbligo di denuncia da parte del possessore. Quindi, uno può possedere un esemplare di pianta tossica nel proprio giardino, che comporta la libera dispersione dei semi, per cui è previsto l'obbligo di distruzione, ma nel contempo non è previsto l'obbligo di denuncia del possesso.

quale queste specie potrebbero proliferare in modo incontrollato, con il rischio di dispersione spontanea o addirittura di introduzione volontaria (perché c'è chi, non volendo denunciare,

e a sospendere l'applicazione delle sanzioni per la mancata iscrizione e versamento dei contributi al sistema di tracciabilità dei rifiuti, fino al subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. del doppio binario si rende necessaria, poiché il Sistri, introdotto nel 2009 e mai entrato in operatività, presenta tuttora rilevanti problemi di applicabilità, in particolare nei confronti delle piccole imprese. Attualmente, dopo aver espletato il bando di gara per un nuovo gestore nell'agosto 2016, non risulta ancora completata e formalizzata la procedura di aggiudicazione e non è stato ancora contrattualizzato il nuovo gestore, anche alla luce dei ricorsi pendenti. Nel frattempo, le apparecchiature sulle quali si basava il vecchio sistema sono ormai obsolete, inefficienti, in disuso e le imprese, non avendo effettuato aggiornamenti e formazione specifica, non sono in condizione di utilizzare il sistema. Inoltre è necessario evitare che nel periodo transitorio, nel quale non è assicurata una corretta e compiuta operatività del sistema, le imprese subiscano pesanti sanzioni per la mancata iscrizione e il connesso versamento dei contributi previsti all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. Si propone pertanto di modificare l'articolo in esame sostituendo la disposizione che prevede il mero dimezzamento delle citate sanzioni con il loro rinvio, almeno fino alla data in cui non subentrerà nella gestione il nuovo concessionario.

e voglio che venga messo agli atti. Chiedo un minuto per illustrare l'emendamento 4.8 che riguarda

l'agevolazione fiscale per gli affitti che avvantaggia sia i locatori, cioè i proprietari di immobili, sia gli affittuari. questo beneficio debba essere prorogato nei termini perché avvantaggia e sicuramente rilancia anche il mercato immobiliare.

affidata al presidente del Consiglio Conte, relativa alla risoluzione della questione Bolkestein che vede coinvolte 30.000 aziende, un milione di persone che lavorano più di 150.000 ambulanti che operano in aree di suolo pubblico. Con questi emendamenti abbiamo cercato di andare incontro a quella risoluzione, approvata da tutti con il parere favorevole del Governo, spostando la questione non più al 2020 ma dando ampia disponibilità e discrezionalità: dieci anni di proroga, oppure trenta, oppure quaranta, oppure sessanta. Insomma, individuiamo un periodo congruo per consentire al Governo di poter lavorare, operare e a tutti noi di fare la nostra proposta e togliere le aziende balneari e gli ambulanti su suolo pubblico dalla problematica della Bolkestein. cosa è successo? In Commissione questi emendamenti, che non hanno nessun riscontro di tipo finanziario né di tipo economico per lo Stato, ma lo hanno per le imprese e per le famiglie, sono stati bocciati. E finché li bocciava il Partito Democratico, come ho detto ieri in Commissione, la cosa non ci sorprendeva affatto. Ma quando a bocciarli sono stati anche i nostri amici e colleghi della Lega, con i quali abbiamo condiviso battaglie, momenti difficili e quant'altro, questo ci ha sinceramente preoccupato. Io vorrei da parte loro, se fosse possibile, un guizzo di riscatto

il Governo e la maggioranza abbiamo perso un'occasione per prorogare la vigenza di un provvedimento che favorisce la locazione a favore delle fasce più deboli della popolazione. Infatti si tratta di prorogare la cedolare secca al 10 per coloro i quali invece di affittare gli immobili a prezzo di mercato, quindi con un lucro certamente maggiore, accettano di affittare a canone concordato, cioè ai canoni che le associazioni e i sindacati rappresentativi degli inquilini concordano insieme agli enti locali per locali per calmierare il mercato. È una misura sociale, una misura che tutela da un lato le classi più povere e disagiate e dall'altro la proprietà edilizia che, in maniera virtuosa, mette i propri immobili anche a disposizione di categorie e fasce sociali più deboli. Da questo punto di vista, voglio sperare che quando andremo alla votazione di questi emendamenti, ci sarà da parte della maggioranza, e forse anche del Governo, un ripensamento rispetto all'opportunità di approvare questa proposta di

Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 4.0.2, che riguarda la possibilità di poter finalmente sbloccare i fondi per le emittenti televisive locali, vicine al territorio, che nel corso degli anni hanno avuto delle difficoltà.

una proroga, ma non posso pensare che il senatore Mallegni, molto esperto, non sappia che le proroghe vengono fatte quando ci sono delle urgenze. Essendo già prorogato al 2020, ci sarà senz'altro l'occasione più giusta per poter procedere in quella direzione. Quindi, la tranquillizzo: la pensiamo alla stessa maniera.

essendo stato presentatore con gli altri colleghi del Partito Democratico di analogo emendamento, poi approvato dalla Commissione con un testo 2. Si tratta di un emendamento molto importante perché consente di evitare consente di evitare un rischio di blocco di fondi per le emittenti locali. Nella scorsa legislatura abbiamo molto operato per una vera e propria rivoluzione, nel senso di una riqualificazione del settore dell'emittenza radiotelevisiva locale, l'introduzione di alcuni parametri meritocratici, che i fondi per tali attività dovessero essere destinati e ripartiti sulla base dell'effettivo servizio di qualità svolto da molte emittenti, in alcuni casi quasi a livello, se non addirittura migliore, del servizio pubblico della RAI. Su questa strada, l'altro giorno, in audizione presso l'8a Commissione, il ministro Di Maio ha per la verità detto di voler continuare, apprezzando il lavoro che il Partito Democratico ha messo in atto nella scorsa legislatura. legislatura. Perché ciò avvenga, adesso bisognerà che nella finanziaria il Governo predisponga un finanziamento congruo del fondo. Ma questo sarà discorso dei prossimi mesi. Nel frattempo, l'emendamento era importante, lo abbiamo presentato, è stato approvato in Commissione e di ciò siamo soddisfatti. Signor Presidente, anche noi ci associamo a quanto già detto da alcuni colleghi intervenuti prima di noi su questo emendamento. Anche noi lo abbiamo presentato a prima firma del La Russa. Questo dovrebbe essere un emendamento condiviso da tutti i Gruppi, perché, da una parte, salva migliaia di posti di lavoro e, dall'altra, incide notevolmente sulla priorità dell'informazione.

4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10,

non votare), si andrebbero semplicemente a prorogare i termini attraverso i quali si potrebbe fare ricorso alla *voluntary disclosure*. Questo vuol dire che daremmo un'opportunità a tutta una serie di connazionali residenti all'estero che non hanno pagato le tasse: mi preme però far rilevare che non si tratta di evasori fiscali, bensì di connazionali che, tratti in inganno dal concetto del divieto della doppia imposizione, spesso, alla luce del fatto che hanno versato le tasse nel proprio luogo di residenza, sono incorsi in errore.

In tempi nei quali, come abbiamo visto oggi, lo *spread* schizza per l'ennesima volta, il fatto che non si approvi un emendamento di questo tipo dimostra purtroppo la pochezza di questo Governo *(Applausi

Prego,

per gli affitti. Il diritto allo studio è l'essenza dell'articolo 3 della nostra Costituzione: significa rimuovere gli ostacoli che impediscono a ognuno di realizzarsi e che, in questo caso, caso, impediscono alle ragazze e ai ragazzi del nostro Paese di essere messi nella condizione di studiare, di essere protagonisti, di diventare classe dirigente, di rivitalizzare anche

a compimento di anni in cui i Governi del Partito Democratico hanno raddoppiato i fondi per il diritto allo studio e hanno introdotto una misura rivoluzionaria, quella della *no tax area* per gli studenti delle famiglie meno abbienti.

abbattere questi muri; muri che voi oggi, signori del Governo, rialzate; sono muri di disuguaglianze, di disparità. Respingendo questo emendamento farete un torto al nostro Paese, un torto signor Presidente, colleghi, contrasteremo con tutta la nostra forza*.

Signor Presidente, è il secondo caso. Sono d'accordo che ci possa essere una repentina trasformazione di un emendamento in ordine del giorno, può anche capitare che i testi non siano pronti, ma sarebbe bene che fossero comunque presentati.

questo tipo di misura nuoccia alla possibilità di venire incontro alle esigenze di salute e di tutela nei confronti dei minori. avvenuto soltanto ieri di due bambini che purtroppo hanno perso la vita deve far riflettere non solo chi propone questo emendamento, ma soprattutto

allo stesso modo, rivolgiamo un accorato invito affinché i proponenti di questo emendamento lo ritirino, perché riteniamo gravemente lesivo degli interessi dei più piccoli, dei minori, prorogare l'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione nelle scuole. Dichiaro pertanto il voto assolutamente contrario del Gruppo Forza Italia.

dell'obbligo, che rimane vigente, ma è un artificio legislativo per consentire di eludere l'obbligo vaccinale (che persiste) ancora per un anno, posticipando la presentazione del certificando di vaccinazione nido e alla scuola materna. È un po' che come se decidessimo di rendere obbligatorie le cinture di sicurezza e poi disponessimo che i vigili non possono fare la multa per un altro anno. Insomma, si tratta un po' di un artificio. un artificio. In realtà il contratto di Governo tra MoVimento 5 Stelle e Lega prevedeva dei provvedimenti, che io auspico, per conciliare la frequenza scolastica con la protezione della salute. In realtà, prorogare di un anno la consegna del certificato vaccinale purtroppo non fa né l'uno né l'altro e oggi c'è stato un appello del presidente del dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità che ha parlato di pericolo per la salute pubblica legato a questo emendamento, pur riconoscendo la libera scelta di questo Parlamento. Esso infatti non tutela né la salute né la frequenza scolastica, ma semplicemente posticipa la consegna del certificato e ciò fa sì che i presidi non conoscano lo stato vaccinale dei bimbi.

di conciliare la frequenza scolastica con la salute. Inoltre questo provvedimento non ha nessuna possibilità di aumentare le coperture vaccinali, come abbiamo sempre dichiarato come MoVimento 5 Stelle. Questo Parlamento è sovrano ed è libero di fare le sue scelte come ha fatto tante volta, su Stamina su tanti provvedimenti su cui avremmo potuto tutelare la salute dei più piccini. Ovviamente io rispetto la scelta del Gruppo cui appartengo e del Parlamento, ma per storia personale, professionale e, dolorosamente, di madre,

ogni scelta politica presuppone una scelta di responsabilità. Qui qualcuno si sta assumendo la responsabilità non di spostare

mettere a rischio la salute non solo dei più piccoli e degli immunodepressi, ma di tutti, perché in questo modo viene meno il senso di comunità. Noi avevamo una linea chiara: insieme all'obbligo, signor Presidente, il decreto Lorenzin

tutta la comunità. Non dimentichiamo che noi siamo qui per tutelare la comunità italiana: facciamolo, perché questo è un servizio che mettiamo a disposizione di tutti. Non assumiamo - anzi, non assumetevi, perché noi voteremo contro l'emendamento in esame - la responsabilità di mettere a repentaglio la salute della popolazione.

la maggioranza ha deciso di votare l'emendamento in esame, che formalmente è un rinvio, ma che dovreste avere il coraggio e l'onestà di chiamare pietra tombale sulla vaccinazione obbligatoria. Avete spesso parlato di onestà, ma l'onestà intellettuale è altrettanto importante di quella di carattere penale e legale. Questo non è un semplice rinvio, ma un rinvio *sine die,* ovvero una pietra

sono mille le volte in cui i provvedimenti vengono rinviati. Quando non si ha il coraggio di dire le cose per come stanno, si preferisce rinviare. Allora, io voglio chiedere

dice che il Parlamento provvederà, perché non si tratta di porre fine alla politica delle vaccinazioni. Allora, se questo è vero, chiedo formalmente a coloro che siedono sui banchi del Governo di esprimersi e di dire che questo è un provvedimento tampone che vale soltanto per qualche mese e che il Governo il Governo e la maggioranza si impegnano a portare in quest'Aula un provvedimento diverso, per la natura e per le finalità, entro la fine di quest'anno. In caso contrario, noi saremo legittimati a pensare quello che ho detto in premessa, ovvero che questa è la vittoria del popolo No Vax, di coloro

non c'è bisogno di una sanzione da parte dello Stato per fare quello che tutti, con buon senso, ritengono necessario. La storia di questo Paese parla,

per tutta la notte il Governo e la maggioranza non dicano una sola parola per giustificare e motivare i loro provvedimenti, non una parola; lo posso capire, perché è un decreto d'urgenza e abbiamo inteso che si legifera a fari spenti. Però su questo tema no: il Governo e la maggioranza dicano cosa pensano e cosa intendono fare.

su una misura coercitiva di un decreto-legge, quello Lorenzin, pasticciato, illiberale e discriminatorio.

ma posticipa di un anno il divieto di accesso al nido e all'infanzia per mancanza di documentazione di avvenuta vaccinazione. Cari colleghi del Partito Democratico, questo emendamento non fa ritornare il Paese nel medioevo, come qualcuno di voi ha detto ieri in Commissione. È un emendamento di buon senso, fatto in assenza dell'istituzione dell'anagrafe vaccinale nazionale, che contempera il diritto alla salute e il diritto all'istruzione individuale e collettiva. Con questo emendamento tutti i bambini della fascia di età tra zero e sei anni a settembre potranno andare a scuola, al nido e all'infanzia.

a scuola i bimbi e gli adolescenti della fascia di età tra i sei e i sedici anni, i quali, secondo il Lorenzin, possono non vaccinarsi, pagare la multa e fermare il virus. Ecco perché è discriminatorio. Per questo motivo il Gruppo della Lega Nord voterà a favore di questo emendamento. senatrice Taverna. Signor Presidente, il mio intervento è per togliere qualunque alibi a chi ha voluto continuare a strumentalizzare una importante forma di prevenzione come quella della vaccinazione che il MoVimento 5 stelle ha sempre sostenuto. *(Applausi dai Gruppo**PD).* L'unica cosa che noi continuiamo a respingere al mittente è la possibilità di voler trattare gli italiani come delle pecore che devono essere obbligate piuttosto che informate. L'unico obiettivo da parte del MoVimento 5 Stelle, che so essere condiviso anche da parte della Lega, è quello di permettere ai genitori che hanno tutte le intenzioni di vaccinare i propri figli di farlo in ambienti che siano in grado di accogliere

dei bambini erano le banche e i finanziamenti

questo significa che, ogni qualvolta viene espressa un'opinione diversa, ci deve essere bagarre? Non è questo il Parlamento! e concludo, non c'è alcun attentato alla salute pubblica, ma c'è un profondo rispetto nei confronti del Paese Italia e dei cittadini italiani che meritano una politica che pensi pensi a loro informandosi e non nascondendosi dietro un obbligo. Stavolta hanno reso obbligatori 10 vaccini ma, considerando come si sono comportati e gli obblighi e le imposizioni cui hanno costretto questo Paese, siamo ben felici di tornare a una Repubblica che sia democratica e consenta a tutti di prendere le proprie scelte in maniera consapevole e di fare il bene del Paese Italia non obbligando, ma informando le persone. È questo quanto si chiede.

questi signori Fuori mando soltanto io. Mandare fuori è una decisione della Presidenza e di nessun altro. Mi auguro che la senatrice Taverna non abbia fatto quel gesto, perché come Vice Presidente ha un ruolo L'abbiamo visto tutti noi e io le dico, Presidente, che non mi permetto di chiedere alla Presidenza di fare ciò che essa stessa può agevolmente decidere. Le devo dire, però, che sono indignato per il fatto che, anche se questi signori ultimamente si vestono di bello, sono sempre i soliti, sempre. *(Applausi dai

di incidere sui rapporti civili ed etico-sociali previsti in particolare dall'articolo 32 Costituzione. Inoltre, secondo la prassi, e comunque anche se fosse ammissibile, le richieste di votazione segreta devono essere presentate in tempo

per le quali è previsto il voto segreto. Dopodiché, se c'è una questione di prassi e di tempo, io le chiedo di accantonare l'emendamento e di porlo in votazione nella prossima seduta, in modo che lei abbia comunque il tempo di informare tutti i colleghi del voto segreto. È una materia così importante, che riguarda la vita dei nostri bambini, che noi non possiamo certo fermarci di fronte a una interpretazione - mi permetta - eccessivamente puntuale e non rispettosa del senso complessivo del tema. Senatore Marcucci, forse non sono riuscita a spiegarmi. Io non ho detto soltanto che c'è una questione di tempi. Ho detto, tra l'altro, che dal mio punto di vista, esiste anche una questione di tempi perché,

come mai c'è stata questa divergenza, perché - altrimenti - l'impressione è di un artificioso modo di parlare, oppure - peggio - che vi sia stato un convincimento, di cui però non abbiamo avuto notizia. In altre parole, la senatrice, che ha manifestato la sua contrarietà all'emendamento,